«La Commissione programmazione-economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.203, 22.201, 22.203, 22.204, 22.205, 23.206, 28.203 e 33.204, nonché, a rettifica del parere già espresso, sulla proposta 1.208. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 23.202 e 24.202. In ordine alle proposte 28.200 e 28.0.200 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che sia specificato che i relativi costi sono a carico dei consigli dell'Ordine. A rettifica del parere già espresso sul testo del provvedimento, in relazione all'articolo 21 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che al comma 2 le parole "del CNF" siano sostituite dalle seguenti: "dal CNF". La medesima condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è altresì resa sulla proposta 21.205. Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti sino all'articolo 33. L'espressione del parere è rinviata su tutti gli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 34, sulla proposta 2.5 (testo 2), nonché su tutti gli ulteriori emendamenti oggetto di riformulazione». «La Commissione programmazione-economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione alle proposte relative all'articolo 34, parere di nulla osta. Il parere è altresì di nulla osta in riferimento alle proposte emendative relative agli articoli 35, 36 e 37. Per quanto riguarda l'articolo 38, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 38.200, mentre in relazione alla proposta 38.700 il parere è favorevole a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia introdotta una clausola di invarianza. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti a tale articolo. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 39, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 39.700, 39.0.200 e 39.0.200 (testo 2), 39.210, 39.211, 39.246, 39.254, 39.266, 39.267, 39.268, 39.269, 39.270, 39.271, 39.272, 39.273 e 39.282. Esprime poi parere di nulla osta sugli emendamenti 39.200, 39.240, 39.244, 39.245, 39.247, 39.248, 39.249, 39.250, 39.251, 39.252, 39.253, 39.255, 39.256, 39.257, 39.258, 39.259, 39.261, 39.274, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia inserito il seguente periodo: "Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito". Infine, in relazione all'emendamento 39.201 il parere è favorevole, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia inserito il seguente comma: "I costi per la costituzione e il funzionamento delle commissioni nonché per l'espletamento delle prove di esame devono essere a carico dei soggetti partecipanti alle prove". In relazione all'articolo 39, il parere resta sospeso sull'emendamento 39.900 e sui relativi subemendamenti, nonché sull'emendamento 39.902. Il parere è di nulla osta sulle proposte emendative riferite all'articolo 40. In relazione poi agli emendamenti riferiti all'articolo 41, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 41.700, mentre è sospeso su tutti i restanti. Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti a partire dall'articolo 42 e sulle ulteriori riformulazioni». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 41.200. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 41.201, 41.202, 41.203, 41.204, 41.205, 41.3 e 41.211. In ordine alla proposta 41.208, il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che alla lettera siano soppresse le parole "e tendenzialmente a carattere gratuito". Il parere è di nulla osta su tutte le altre proposte emendative riferite sino all'articolo 45. Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti a partire dall'articolo 46 e sulle ulteriori riformulazioni». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti a partire dall'articolo 50, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 50.207, sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 50.202 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione del seguente periodo: "I componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le trasferte effettuate in adempimento di ogni compito loro affidato". In relazione agli emendamenti 64.700 e 66.0.700 il parere è altresì di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la parola: "possono" sia sostituita dalla parola: "devono". Il parere è sospeso sugli emendamenti 2.5 (testo 2),

20.900 e relativi subemendamenti, 22.700, 28.700, 39.900 e relativi subemendamenti, 39.902, 46.900 e relativi subemendamenti, 13.200 (testo 2), 10.0.200 (testo 2) e 10.232 rinviato dall'Assemblea in Commissione».

Presidente, credo sia opportuno intervenire sull'ordine dei lavori prima di riaprire la discussione in Aula sul provvedimento di riforma dell'ordinamento forense. Come i colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta - l'ultima nella quale ci siamo occupati di questo testo - si era presa la decisione, a nostro avviso saggia, e condivisa dal presidente Schifani, di riportare il testo in Commissione perché

La Commissione, purtroppo, non è servita in alcun modo a dipanare tali questioni, né ad approfondirle - mi permetto di dire fuori dai denti - e neanche ad ascoltare le ragioni dell'opposizione o di coloro i quali comunque sono critici nei confronti di questo provvedimento, né a trovare una soluzione condivisa o a spiegare le ragioni per le quali alcune posizioni vengono sostenute in maniera così recisa.

pregiudiziale per il Gruppo del Partito Democratico), la cancellazione dall'albo (abbiamo avuto una surreale discussione sul fatto che non si è riusciti neanche ad approvare la norma che prevede che non possano essere più iscritti all'albo gli avvocati che abbiano riportato una sentenza di condanna passata in giudicato per reati

sia pure con soluzioni diverse, accenti unanimi in tutto il Parlamento italiano). Queste cinque questioni, essenziali per ridisegnare la professione dell'avvocato e consentire l'apertura del mercato di questa professione liberale ai giovani professionisti, sono state oggetto di una chiusura assoluta da parte della maggioranza. Torniamo in Aula con le stesse rigidità di prima e, purtroppo, in un clima politico che non solo non è rasserenato ma trova

maggioranza, anche di fronte alle interessantissime prese di posizioni che sono venute in quest'ultimo periodo dalla Confindustria e senza volere in nessun modo rallentare un *iter* che probabilmente è anche giusto trovi il suo esito prima del congresso nazionale del CNF; insomma, è una questione essenziale per ridisegnare il profilo della competitività dell'Italia e mi chiedo se sia questo il modo per affrontarla. Ciò, tra l'altro, pone un'ulteriore questione, cui accenno soltanto perché non voglio rubare più tempo all'Aula. Le Commissioni del Senato e probabilmente le Commissioni parlamentari non riescono più ad essere, anche in ragione dell'organizzazione dei lavori che dedica troppo poco tempo alle stesse, il luogo di un'istruzione dei provvedimenti che possa sfuggire all'animosità, che è normale si sviluppi nell'Aula, e veda invece i propri lavori affidati alle qualità di competenza, capacità di approfondimento e rispetto delle posizioni reciproche tra i diversi Gruppi rappresentati in Parlamento.

È da tantissimo tempo che la nostra Commissione, prima in Comitato ristretto e poi in sede plenaria, ha affrontato un confronto serrato e costruttivo tra opposizioni e maggioranza.

Poi c'è stato un cambiamento di opinione da parte delle opposizioni, o perlomeno da parte del Partito Democratico (perché l'Italia dei Valori si è distinta dal Partito Democratico):

per altro verso, si trattava di emendamenti che erano in evidente contrasto con la filosofia che aveva ispirato questo disegno di legge,

Ma è mai possibile, onorevole Presidente, fare una riforma dell'ordinamento professionale forense disinteressandosi dalle attese degli avvocati italiani, dalle aspettative dei 230.000 avvocati italiani? che il collega Ichino è portatore di una filosofia completamente diversa da quella che ha ispirato la maggioranza, ma mi rendo anche conto che

per associarmi alle considerazioni svolte dalla presidente Finocchiaro. Dando atto al presidente Berselli di aver fatto di tutto per cercare di mediare,

la situazione è stata esattamente questa. Rinviata questa normativa alla Commissione, si è discusso a lungo sui primi articoli, per poi renderci conto che non vi era possibilità di mediazione. Il presidente Berselli ha proposto all'opposizione Il presidente Berselli ha proposto all'opposizione di portare alla discussione qualche punto, sul quale vi era intransigenza e dal quale non si poteva prescindere. Pertanto, d'intesa con l'altra parte dello schieramento, cioè il Partito Democratico e l'Italia dei Valori, abbiamo raggiunto un accordo su cinque punti. Questi cinque punti prevedevano un'apertura verso i giovani.

fare in modo che chi fosse condannato per mafia e terrorismo non potesse essere iscritto all'ordine degli avvocati. Non c'è stata possibilità di discutere alcun punto.

evitare una riforma che ci allontani dall'Europa e che, di fatto, penalizzi, non tanto e non solo l'accesso delle giovani generazioni

di continuare ad esercitare in modo compiuto la loro attività. Per questo motivo, noi avremmo preferito un confronto

l'emendamento 17.214 è precluso. In queste condizioni la Presidenza è dell'avviso di accantonare l'articolo 17, per mancanza dei pareri,

siano assolutamente contraddittori tra loro e provengano dall'approvazione in Aula di testi su cui il relatore ha dato parere favorevole

si è stabilito che l'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza svolge le attività di cui ai commi 5 e 6. È stato cioè eliminato il riferimento alle parole «in via abituale e prevalente». Successivamente, all'articolo 20, l'emendamento presentato dal relatore in Commissione va in direzione totalmente opposta. Questo sistema basato sugli accantonamenti, per cui non si capisce più la logica di un provvedimento, rende rende impossibile ottenere un testo decente, signora Presidente. Questo Parlamento è pieno di giuristi. Noi ci dobbiamo vergognare per i testi che licenziamo; non riusciamo infatti a spiegare all'opinione pubblica perché siano così incoerenti e contradditori.

favorire un accordo su determinati punti qualificanti. Ho chiesto più volte al presidente Berselli di informare il Presidente del Senato del fatto che non era possibile raggiungere un accordo, certo non per mancanza di una volontà costruttiva da parte delle opposizioni.

allora come sia possibile proseguire in questo modo. Io la prego, signora Presidente, di voler sinceramente rimettere in discussione la possibilità di andare avanti.

Il filo logico c'è; ma, se andiamo avanti con questo sistema incoerente, non potremo raggiungere alcun risultato positivo. Da ciò è chiaro ed evidente che

Presidente, io credo che si debba seguire il criterio che è sempre stato adottato, proseguendo con

Ritornare indietro significherebbe infatti ricominciare da capo. Noi abbiamo già le idee chiare. Quelli accantonati sono emendamenti sui quali si è fatta una riflessione puntuale anche in Commissione:

non si è trovata una sintesi e non si è trovato un accordo. Ognuno ha proposto e difeso le proprie ragioni, nella piena consapevolezza che esse dovessero prevalere.

e valutarle nella forma più consona. Credo si debba seguire l'ordine dei lavori com'è stato finora condotto.

18, la cui trattazione si era interrotta quando fu deciso di assumere le determinazioni note.

solo far osservare che abbiamo accantonato l'articolo 17, che tratta la materia delle incompatibilità, l'articolo 18 ha come oggetto le eccezioni alle norme sulle incompatibilità. Qualcuno può spiegarci come sia possibile discutere delle eccezioni se non sappiamo ancora quali sono le norme generali sulle incompatibilità? Questo è solo un esempio, perché potremmo farne altri dieci. Gli articoli che abbiamo accantonato stabiliscono principi generali della materia. Più si va avanti e più si va nel dettaglio. Non è materialmente possibile e non ha alcun senso logico procedere nella discussione,

i primi 16 articoli. Poi c'è l'accantonamento di tutti gli emendamenti che riguardano l'articolo 17

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.5 (testo 2), 8.223 (testo 2), 10.0.200 (testo 2), 10.232, 8.230 (testo 3)/6 e 21.205 e relativi subemendamenti. Sull'emendamento 13.200 (testo 2) il parere è di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 6 siano aggiunte le parole: "fermi restando gli obblighi contributivi vigenti". Sull'emendamento 39.902 il parere è di nulla osta, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia soppresso l'ultimo periodo del comma 2 e sull'emendamento 8.230 (testo 3) a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, dopo la parola: "stabilisce" siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 22.201 (testo 2), 22.700 (testo corretto), 28.700 (testo corretto), 24.202 (testo 28.0.200 (testo 2), 28.0.200 (testo 2)/l e 28.0.200 (testo

46.900, 47.1000/2, 64.700, 66.0.700, 2.218 (testo 3), Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo d'Aula n. 3».

la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questo pomeriggio, ha approvato modifiche al calendario corrente ed il nuovo calendario dei lavori fino all'11 novembre 2010. Le sedute di questa settimana sono dedicate al seguito dell'esame del disegno di legge di riforma della professione forense. Nella giornata di giovedì 4 novembre i lavori dell'Assemblea si concluderanno alle ore 12, su richiesta del Gruppo del Popolo della Libertà in relazione ad un impegno politico. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 16, in occasione della ricorrenza del 4 novembre, si svolgerà nell'Aula del Senato un evento in commemorazione dei caduti della Brigata Julia in Afghanistan, con l'esibizione di quattro cori alpini. Nella seduta pomeridiana di martedì 9 novembre, il Ministro dell'interno renderà un'informativa su questioni che hanno riguardato la questura di Milano. Successivamente interverranno i rappresentanti dei Gruppi. In relazione alla disponibilità del Ministro l'informativa potrebbe essere anticipata

di una sua possibile conclusione entro la giornata di mercoledì 10 novembre. *(Commenti dal Gruppo PD).* A tal fine i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi secondo criteri non proporzionali

sull'esecuzione domiciliare di pene detentive, ove non riassegnato in sede deliberante. Nel corso della prossima settimana saranno inoltre discusse la mozione Ghedini su benefici a favore di vittime del terrorismo e la mozione Li Gotti sulle candidature elettorali nelle elezioni regionali amministrative, nonché ratifiche di accordi internazionali. In occasione della prossima Conferenza dei Capigruppo, da convocare nella giornata di martedì 9 novembre, saranno calendarizzati il seguito della mozione Rutelli, D'Alia, Pistorio sulla politica economica e la mozione Baio sulla patologia della depressione.

coloro che mi hanno proposto di rinviarne la valutazione in quella sede hanno puntato semplicemente a una dilazione ingannatoria. Credo che non si tratti di questo, ma di una dimenticanza, per quanto spiacevole,

i suoi documenti per quanto riguarda le politiche economiche) prima che il Governo si pronunci rispetto all'Europa, sarebbe non solo corretto con l'impegno preso, ma anche ragionevole in relazione a quanto accade nel Paese e rispetto a ciò che di surreale accade nell'Aula del Senato della Repubblica a proposito della riforma della professione forense. Quest'ultima forse si concluderà la settimana prossima, ma non escludiamo la successiva, per finire magari su un binario morto nelle settimane ancora successive. Chiedo scusa per una certa mia animazione, che non è offensiva verso il presidente Azzollini, ma mi auguro che si trovi un'intesa.

È verissimo che il presidente Gasparri, in sede di Conferenza dei Capigruppo, ha posto la questione. Se mi posso permettere di anticipare per le vie brevi quanto ho appena appreso dal Segretario generale,

segue: «la maggioranza assume l'impegno di richiederne alla Conferenza dei Capigruppo la calendarizzazione per il giorno 9 vorrei rappresentare all'Assemblea, e in particolare al senatore Rutelli - la presidente Bonino era presente ai lavori della Capigruppo - che è stato il sottoscritto - collega Rutelli - a porre il problema della calendarizzazione

Si può discutere di tutto, ma, come la presidente Finocchiaro annuendo conferma... Questo lo dico sul piano dei rapporti di Aula, senatore Rutelli, a cui tengo. Dopodiché, il problema è il

Non so quando potremo farlo, ma mi auguro che si possa aiutare l'Europa a risolvere al meglio i suoi problemi anche attraverso la mozione della quale io ho chiesto la discussione. Decida la Presidenza, a questo punto, che cosa fare.

l'unanimità in questa sede - già a partire da martedì 9, se l'Assemblea lo ritiene, evidentemente dopo l'informativa del ministro Maroni, qualora l'informativa avvenga martedì e non

della questione, a meno che, evidentemente, la prossima Conferenza dei Capigruppo, che comunque sarà convocata nella giornata di martedì, decida oltremodo. Altrimenti, rimane il calendario attuale, con l'inserimento, all'unanimità, della mozione Rutelli ed altri.

è assolutamente corretto quello che si sta per decidere, se ho capito bene, all'unanimità: cioè che si discuta o il 9 o al più tardi il 10 mattina la mozione Rutelli. Ricordo, solo per precisione, che nella risoluzione che abbiamo approvato alla fine del dibattito della scorsa settimana vi è un impegno del Governo, che ovviamente dovrà essere soddisfatto nella stessa circostanza, a presentare entro il 10 novembre - scritto così nella risoluzione - in Parlamento la bozza del Piano nazionale per le riforme. Intendo che la decisione di calendarizzare la mozione Rutelli, assolutamente coerente con questo punto all'ordine del giorno, riguardi anche il fatto che in quella occasione il Governo riferirà sul Piano nazionale delle riforme.

che il Consiglio dei ministri della scorsa settimana ha discusso il Piano nazionale delle riforme, e quindi penso che il Governo sia perfettamente attrezzato a presentarsi in Parlamento la prossima settimana con questa bozza.

Colleghi, come avete tutti sentito, il parere della Commissione bilancio, piuttosto consistente, è appena arrivato. Bisogna dare il tempo agli Uffici, nonché ai colleghi,

ricordo - è notizia di queste ore - che è stata probabilmente decretata la condanna a morte di Sakineh Ashtiani e che i rappresentanti di vari Gruppi hanno depositato una mozione al riguardo. Due settimane Due settimane fa alla Camera dei deputati è stata discussa una mozione simile, che si è ampliata anche con riferimento alla campagna, che l'Italia guida nel mondo, per la risoluzione sulla moratoria universale della pena di morte. Da allora ad oggi sono occorsi ulteriori gravissimi fatti relativamente ad alcuni familiari di Sakineh Ashtiani

la votazione è chiusa.

a chi non è iscritto all'albo degli avvocati l'esercizio della consulenza in materia legale (parliamo ovviamente di consulenza stragiudiziale). Noi non possiamo procedere su questo terreno se non considerando attentamente il fatto che le nostre università sfornano ogni anno decine di migliaia di laureati in giurisprudenza, dei quali meno del 10 per cento si iscriverà a un albo degli avvocati; tutti gli altri sono destinati a esercitare le loro conoscenze giuridiche al di fuori della professione forense.

Tutti i laureati di queste altre facoltà si vedrebbero inibita la possibilità di esercitare le proprie conoscenze giuridiche in un rapporto professionale,

arrivo a dire - anche incostituzionale, perché è evidente che non c'è alcuna ragione di carattere economico o sociale per questa limitazione, se non quella di creare una rendita di posizione per il ceto forense. Datemi un solo motivo per cui debba essere vietato a un laureato in scienze politiche, in economia o in legge, che non sia iscritto all'albo, di esercitare le proprie conoscenze giuridiche nel proprio lavoro, anche a vantaggio di un cliente o di un committente con il quale abbia instaurato un rapporto professionale: se non mi sapete dare una ragione per questo, dovete riconoscere che questa norma, non avendo ragion d'essere, è irragionevole e incostituzionale.

se proprio volete che questa norma venga approvata, almeno formulatela in un modo tecnicamente accettabile. all'albo esercitare le proprie competenze giuridiche soltanto in favore del datore di lavoro, purché sia esclusivamente nel suo interesse, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato oppure di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

al contratto di società con il lavoro come conferimento personale, al lavoro in partecipazione, al lavoro cooperativo,

il giudizio del senatore Ichino, nel senso di ritenere che questo sia uno dei passaggi più significativi del disegno di legge Noi, come Gruppo dell'Italia dei Valori riteniamo che la consulenza legale debba essere riservata a chi abbia il titolo per renderla. Senatore

di un atto di querela, che non è un atto del giudizio, ma di impulso al giudizio, che venga redatto non da un

La querela non è un atto giudiziale, senatore Ichino, bensì un atto stragiudiziale, perché introduce: è una richiesta di giudizio. Mi dispiace doverla contraddire. La querela, pur se ne

richiedo; è un'invocazione di giudizio, non è un atto giudiziale. Affidato alla gestione di chi non sia avvocato, e che quindi non si assume la responsabilità di ciò che va a compiere il querelante, è un atto, questo sì, di irresponsabilità,

Senatore Casoli, vada al suo posto, per favore. Proprio lei che dovrebbe collaborare nel regolamentare i lavori d'Aula!

Colleghi, per favore, ciascuno al proprio posto.